vi informo che la Conferenza dei Capigruppo è stata temporaneamente sospesa e riprenderà alle ore 10,15. Abbiamo mezz'ora di tempo per affrontare un tema che considero molto rilevante e che la Conferenza dei Capigruppo ha autorizzato a trattare subito, in apertura di seduta, ovvero la crisi politica in Venezuela.

affettuoso e sincero, spero rappresentativo di tutto il Parlamento, agli italiani che vivono in Venezuela *(Applausi)* e che in questo momento soffrono pesantemente le conseguenze di una situazione che si protrae da diversi anni. Onorevoli colleghi, credo che tutti abbiamo assistito con apprensione a quello che sta accadendo in Venezuela. Vorrei dire una cosa in premessa. Sul Venezuela la politica italiana negli anni passati si è divisa pesantemente: del Venezuela abbiamo dato giudizi diversi; storicamente del chavismo sono stati dati giudizi diversi. Ma oggi non è il momento di riaprire la pagina delle discussioni storico-politiche. Oggi è il momento di guardare in faccia la realtà e di vedere come uno dei Paesi che negli anni Settanta era tra i più ricchi del mondo, ai vertici di tutte le statistiche mondiali, oggi si è ridotto ad essere un Paese in cui un decimo della popolazione è scappato, il 90 per cento vive sotto i livelli di dignità,

il cibo razionato; la produzione petrolifera è scesa da 3 milioni di barili a 900.000 e, probabilmente, nei prossimi mesi si arresterà, per la semplice ragione che non sono state adeguate le attrezzature in tutti questi anni, e quindi anche l'unica risorsa di cui il Paese dispone si sta inaridendo. Davanti a questa situazione, colleghi, sapete benissimo che negli anni scorsi sono intervenute le autorità internazionali, dall'ONU all'Organizzazione degli Stati americani, dal Mercosur a quella che è la principale risorsa spirituale del Venezuela, la Chiesa cattolica con la Conferenza episcopale. Non solo. Il Santo Padre, Papa Francesco, e il Vaticano sono intervenuti più volte anche per cercare di proporsi - poiché avevano il consenso di tutti, del regime e dell'opposizione - come elemento di dialogo politico. Ricordo ai colleghi - molti di voi

che i nostri connazionali volevano medicinali; alcuni nostri funzionari dell'ambasciata avevano avuto congiunti morti per malattie abbastanza banali e non c'erano medicinali. Ma davanti alla richiesta delle autorità italiane di fare arrivare i medicinali alla nostra comunità, il Ministro degli esteri venezuelano aveva detto al nostro Ministro degli esteri che in Venezuela le cose andavano bene,

dei medicinali e delle persone bisognose. Ebbene, tutto questo naturalmente non ha prodotto nulla, perché era una scusa per non accettare medicinali dall'estero. Vi dico di più. C'è stata la proposta della Chiesa di ergersi a mediatrice, ma si chiedeva la liberazione dei prigionieri politici e il ripristino delle tappe tappe elettorali, le elezioni liberamente convocate. Ebbene, tutto questo ha prodotto un muro di diniego, al punto che il Santo Padre e la Chiesa cattolica si sono ritirati rispetto a qualsiasi ipotesi di lavoro, perché non c'era la possibilità In questi ultimi giorni la situazione è degenerata: è stata costituita un'Assemblea costituente priva di basi giuridiche pur di mettere una "zeppa". A cosa,

istituzione venezuelana legittimata democraticamente è il Parlamento di quel Paese. Cosa è stato fatto, dunque, al Parlamento venezuelano? I parlamentari sono stati privati dello stipendio

tutti questi Paesi, compreso il Canada, hanno riconosciuto la legittimità istituzionale e politica non di chi si è autoproclamato Presidente dello Stato, ma di chi semplicemente

Presidente, questo non è un momento qualunque nei rapporti tra l'Italia e il Venezuela e non è uno dei tanti dibattiti che si sono svolti nei mesi e negli anni passati. Prima il presidente Casini diceva giustamente che nel passato, anche recente, il nostro comportamento è stato diverso nei confronti del Venezuela e del suo Governo. Io stesso, nel mio mandato di Governo, pur non avendo alcuna simpatia per i Governi politici di Chavez e poi di Maduro, sono stato in missione ufficiale in Venezuela, per tutelare la rappresentanza della comunità italiana e per tutelare le imprese italiane, e ho incontrato l'allora presidente Chavez, come tanti tra noi. Un rapporto giusto e legittimo tra le istituzioni di Stati liberamente riconosciuti e i loro Governi liberamente eletti. Ma qui è un'altra storia. Maduro è stato eletto con un plebiscito non riconosciuto dalla comunità internazionale, un anno fa. È un usurpatore, mentre il presidente Guaidó è espressione dell'unico Parlamento eletto liberamente e costituzionalmente dai cittadini venezuelani; egli, sulla base di un articolo della Costituzione venezuelana (il 233), ha assunto la Presidenza, destituendo l'usurpatore. Il Governo legittimo, secondo la stessa Costituzione venezuelana e secondo tutta la comunità internazionale, è quello che Guaidó Guaidó ha espresso ieri, come espressione dell'unico Parlamento eletto. Nello scorso anno, per aggiungere qualche elemento a questa Assemblea, milioni di venezuelani hanno attraversato il confine con la Colombia e con altri Paesi confinanti, per potersi nutrire, per potersi nutrire, curare, acquistare medicine e poi rientrare nel proprio Paese. Ripeto, venti milioni di persone hanno attraversato il confine per poter sopperire alle proprie necessità di sopravvivenza, anche sanitaria. La mortalità infantile è aumentata del 30 per cento. Un milione di venezuelani sono già nei campi profughi all'estero. Il crollo dell'economia venezuelana, una volta florida, è evidente a tutti. La povertà ormai riguarda tre quarti della popolazione non riesce a nutrirsi a sufficienza e un abitante su tre non riesce a mangiare tutti i giorni. La situazione è drammatica. Di fronte a questa situazione drammatica, l'evento di ieri è una svolta. Ma noi dobbiamo essere tempestivi (lo dico al Parlamento e al Governo): se l'Italia interviene riconoscendo il Governo legittimo di Guaidó facendo capire all'usurpatore e, soprattutto all'esercito venezuelano, che un'eventuale repressione sanguinosa (come potrebbe verificarsi nelle prossime ore, se noi restassimo silenti)

di essere portati davanti al tribunale internazionale per crimini contro l'umanità, la repressione non ci sarà. Il nuovo Governo ha già garantito (il presidente Guaidó è stato intelligente in tal senso) l'amnistia per qualunque uomo militare in divisa, qualunque crimine abbia commesso nel passato, purché si schieri con il Governo legittimo, cioè con quello dell'Assemblea nazionale elettiva. Siamo a un momento di svolta che la comunità internazionale si comporti come hanno fatto ieri praticamente quasi tutti gli Stati dell'America meridionale. È emblematico e significativo che, qualunque sia stato e qualunque sia il Governo degli Stati dell'America meridionale, si siano schierati tutti il Governo legittimo di Guaidó e contro ogni repressione. Se anche l'Europa lo farà (come noi ci auguriamo) - e l'Europa è l'America latina, per cui è più importante quello che sceglie l'Europa piuttosto che quello che sceglie il Canada per l'America Latina

che la comunità internazionale non perdonerà mai coloro che dovessero schierarsi per la repressione interna. Questo è importante; in questo momento la diplomazia e la cautela di coloro che dicono di aspettare ancora favoriscono in qualche misura misura la repressione. In questo momento il silenzio è complicità di quello che accadrà. Dobbiamo saperlo e soprattutto lo sanno i 2 milioni di oriundi italiani che vivono e soffrono in Venezuela. Non possiamo lasciarli soli. Chiediamo al Parlamento, al Senato in questo momento e, tramite la Presidenza del Senato, al Governo italiano, di dichiarare immediatamente il riconoscimento del Governo di Guaidó. Senza se e senza ma tutte le forze politiche in questo Parlamento devono dichiararsi e schierarsi. Chi tace favorisce la repressione e porta con sé, nella sua coscienza, anche quello che accadrà.

Signor Presidente, le ultime notizie che arrivano dal Venezuela non sono certo incoraggianti, per usare un eufemismo; parlano di 14 morti e di 218 arresti. Si tratta però solamente del primo bilancio, purtroppo annunciato nelle scorse settimane. Era chiaro che con il giuramento di Maduro le provocazioni rispetto a quella che non è l'opposizione, ma che ha vinto le elezioni ed è legittimata dal punto di vista parlamentare, parlamentare, ci fossero delle manifestazioni che chiedessero di rispettare l'esito parlamentare e denunciassero quanto era accaduto con le elezioni di Maduro. La reazione dei Paesi europei e dell'Unione europea è stata blanda.

È chiaro infatti che il bilancio di cui parlavo prima può aumentare. I dittatori sono soliti fare delle prove per capire che spazi hanno nella loro reazione, che può essere sanguinaria. È evidente che è il momento di dire da che parte si sta. Ho apprezzato le parole di un avversario politico, che oggi è Presidente del Parlamento europeo, che con coraggio nei giorni scorsi ha denunciato con forza

I Paesi dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) lo hanno fatto con estrema velocità, anche maggiore rispetto al passato. Si sa che in quei Paesi è molto importante capire cosa fanno le forze di polizia e che cosa fa l'esercito. Sono altresì sensibili a capire

ma oggi è il momento di decidere se si sta dalla parte della libertà o dalla parte della repressione.*(Applausi dal Gruppo PD)*. E stare dalla parte della libertà vuol dire dare con forza il nostro sostegno al presidente dell'Assemblea nazionale Guaidó. Da questo punto di vista penso che anche il Senato possa far sentire la propria voce e chiedere al Governo di intervenire tempestivamente per mettere in campo tutte le iniziative per garantire la sicurezza della nostra comunità italiana presente in Venezuela ma, allo stesso tempo, per dare un segnale politico qui, dentro l'Assemblea, perché il Governo lo dia all'Unione europea. L'Unione europea non può restare neutrale e deve dire anche lei che sta dalla parte dei princìpi e dei valori che sono iscritti nella Costituzione e nei trattati europei. Per questo noi chiediamo

Signor Presidente, da anni il Venezuela sta attraversando una grave crisi economica, umanitaria e politica; da ieri rischia anche di andare incontro a un conflitto civile, con effetti devastanti che sarebbero pagati dal popolo. Il regime di Nicolas Maduro è da tempo in guerra contro il suo popolo, cancellando tutti i diritti democratici. I venezuelani soffrono la fame per l'iper-inflazione e, come se non bastasse, ogni giorno, da mesi, muoiono persone per mancanza di cure mediche: non soltanto perché è stato smantellato il sistema sanitario nazionale, ma anche per la mancanza di attrezzature e medicine. cento dei bambini è a rischio di morte per la malnutrizione acuta. La violenza è allarmante. Non solo la criminalità organizzata è sotto controllo, ma la repressione governativa è sempre più violenta: si parla di oltre settemila casi di tortura, oltre settemila processi per dissidenza. Vorremmo inoltre ricordare che il Venezuela accoglie la terza comunità italiana in ordine di importanza in tutto il Sudamerica e, se si calcolano i discendenti, parliamo di oltre due milioni di persone. Il Governo italiano deve far sentire la sua voce e prestare immediatamente soccorso ai connazionali in pericolo. Chiedo, anche per questo, che il Senato costituisca da subito il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, già costituito dalla Camera dei deputati. Nonostante una delle componenti politiche del Governo abbia fatto mesi fa un sorprendente *endorsement* verso il dittatore Maduro, Forza Italia sarà sempre dalla parte di chi soffre per la privazione delle libertà. Nonostante questo, un Paese serio non si divide sulla politica estera. Facciamo, maggioranza e opposizione, un appello congiunto al dialogo per evitare la guerra civile e chiediamo a gran voce che in quel Paese si ripristinino immediatamente i diritti democratici e i diritti umani. Sappia, il popolo venezuelano che l'Italia sarà sempre al suo fianco. *Que viva* *Venezuela!*

*(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio i nostri Capigruppo per avere inserito questo argomento in questo argomento in questo momento di pausa (e che pausa, abbiamo visto, non è). Ovviamente anche il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni del Venezuela tutto e, in particolare, ai nostri concittadini che sono o residenti all'estero oppure che si trovano lì in questo momento per

È chiaro che questo è un momento importante per l'Italia e il Governo del cambiamento ha dato un segnale importante, anche e soprattutto in politica estera. Ritengo di parlare a nome di tutta la maggioranza e possiamo ribadire il concetto che il Governo del cambiamento ha dato un segnale di cambiamento anche in politica estera e, soprattutto, con posizioni

la Farnesina, non più tardi di tre giorni fa (quindi senza nessuna presa di posizione o, come si suol dire, senza mettere le mani avanti), ha stipulato un accordo con il Governo venezuelano per la messa a disposizione dei cittadini italiani di medicinali, quelli che avete menzionato questa mattina. *(Applausi dal

e questo il Governo italiano ha fatto. Che cosa vuole di più?

LUCIDI *(M5S)*. Purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesima constatazione della situazione del Sudamerica, che per troppi anni è stato dimenticato: ce ne ricordiamo soltanto quando accadono episodi di questo tipo. Sicuramente sarà il momento per riaprire un grande dibattito parlamentare su come intervenire anche

italiani all'estero e quindi sarà questo il momento anche per approfondire questo tema in maniera molto più concreta e - ripeto - urgente. Sinceramente non ho capito quali sono le motivazioni di questo disappunto perché, secondo me, stiamo lavorando in maniera assolutamente unanime e condivisa. Quindi, tutte queste polemiche sinceramente non le

capire cosa ha fatto il nostro alto rappresentante per gli affari esteri nell'Unione europea nei confronti di questo argomento. Prima di fare tante polemiche, cominciate a farvi un esame di coscienza. *(Commenti del senatore Urso)*. Venite qui a raccontarci cosa avete fatto prima di contestare il Governo del cambiamento che, come vi ho raccontato, anche se non avete voluto ascoltare, sta iniziando a dare dei segnali e a portare degli elementi concreti di cambiamento anche per quelle popolazioni e per quei cittadini cittadini italiani che da troppo tempo stanno chiedendo aiuto.

se non con un'espressione di grande vicinanza, prima di tutto agli italiani in Venezuela ma anche a tutti i venezuelani che in questo momento stanno soffrendo per le vicende che voi tutti avete illustrato.

La Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi nelle fasi di discussione che non prevedano votazioni. Il calendario della settimana dal 5 al 7 febbraio potrà essere integrato con una informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti eventi della politica internazionale, come richiesto nel dibattito che si è svolto in

del decreto-legge sulle semplificazioni. A questo punto il lavoro è rinviato alla settimana prossima; ne prendiamo atto sottolineando che ciò è stato determinato unicamente da questioni interne alla maggioranza e non certo da un atteggiamento non collaborativo da parte delle opposizioni, che invece hanno lavorato con la massima collaborazione. Per la verità, hanno lavorato anche con la collaborazione da parte della maggioranza in Commissione. Tuttavia, per problemi

o di partecipare con i suoi membri ai lavori d'Assemblea, senza stravolgere i tempi di approvazione del decreto-legge sulle semplificazioni. Se però

importante nonché sui recenti accadimenti in Venezuela. Il ministro Moavero Milanesi, come tutto il Governo, deve comprendere che il Parlamento è parte

quando abbiamo chiesto al Governo di sapere con certezza se il provvedimento sarebbe arrivato o no in Aula. Il risultato è stato un rinvio continuo e lasciatemi

A fronte di questo, però, c'è stato un problema politico di cui non si parla più. Non nascondiamoci dietro a un dito: i lavori della Commissione sono andati avanti tra *stop and go*, mentre un Ministro ha minacciato di dimettersi e sulla stampa a un certo punto

C'è stato un problema politico all'interno di questa maggioranza e non è un caso che in Commissione la maggioranza continui a presentare emendamenti a se stessa. In genere sono le opposizioni che presentano gli emendamenti e non la maggioranza, che ne ha presentati una montagna. C'è stato un problema politico

questo calendario dei lavori, per attirare l'attenzione su un metodo che respingiamo. Come ieri ha detto anche il nostro capogruppo Ciriani, la pazienza è finita. Noi vogliamo lavorare e vogliamo farlo bene. Abbiamo avanzato la controproposta di continuare a lavorare fino a domani e poi ricominciare martedì. È stato inteso dare un altro calendario: ne prendiamo atto, ma voteremo contro per le ragioni che ho appena enunciato e perché è veramente

dovranno essere presentati nel termine di due ore lavorative dal momento della trasmissione dei testi ai Gruppi. Ciò vuol dire che, se il testo viene trasmesso alle ore

Io sollecito il Governo del cambiamento a darsi un po' da fare e a non tenere in ostaggio l'Aula per un paio di giorni, senza che succeda nulla. È questa una perdita di tempo per tutti noi. *(Applausi dal

intervengo solo per dire che non è vero quello che state dicendo. Abbiamo solo detto che non possiamo né oggi,

Capisco l'intervento del collega Capogruppo della Lega, ma la verità è evidente. Noi abbiamo chiesto ieri di sentire il ministro Moavero Milanesi sul tema rilevante dei rapporti internazionali all'interno

Proprio perché la maggioranza e il Governo si stanno, con costanza, rifiutando di portare in quest'Aula il tema della politica estera scellerata che la maggioranza e il Governo stanno conducendo in Europa e fuori dall'Europa, noi siamo d'accordo affinché il ministro Moavero Milanesi venga il prima possibile a riferirci

Noi lo vogliamo sapere! Il Senato ha il diritto di saperlo! Il Governo ha il dovere di venire a riferire al Parlamento! Ha il dovere! *(Applausi questo che capisco essere, con il loro modo di fare, un ingombro. Per noi il Parlamento non è un ingombro. Il Parlamento è il luogo dove la democrazia

la stimo e capisco benissimo che lei, naturalmente, fa la parte sua. Capisco anche che su un provvedimento come quello in discussione ci possano essere questioni di maggioranza, perché non sarebbero le prime

c'è una questione diversa. Qui c'è una questione di attualità politica su cui noi chiediamo che il Governo venga a riferire. È una cosa che tradizionalmente non si è mai negata.

abbiamo in questo momento deciso in Conferenza dei Capigruppo di dare, su richiesta delle minoranze, tutto il tempo necessario in Commissione per poter lavorare sul decreto-legge semplificazioni. Se la Commissione è convocata e deve lavorare per il decreto semplificazione oggi

per un'informativa, che era poi l'idea originaria. Questa è la proposta che avanziamo e che vogliamo venga messa ai voti.

stare adesso. MALAN *(FI-BP)*. Non lascio stare, perché ci sono dei lavoratori qui. Noi non siamo considerati tali, ma ci sono delle persone che hanno diritto alla tutela della sicurezza sul posto di lavoro e non può esserci costantemente in quest'Aula un volume superiore a quello consentito nei posti di lavoro, incluse le officine meccaniche.

due concezioni della politica estera. Chiunque ha un minimo di cognizione di cosa sia la politica estera, sa che il tempo in questo caso ha una geometria variabile. Voglio dire che, mentre un decreto-legge può essere votato oggi o la settimana prossima, in politica estera ci sono eventi che avvengono in alcune fasi e addirittura

ben chiara e basta che ognuno di noi lo sappia: vuol dire che quella materia è considerata un problema che viene dopo i nostri affari interni e non vogliamo intervenire nel momento nel quale il problema si definisce. Un colpo di Stato o una situazione di difficoltà, se presi in considerazione dopo tre o quattro giorni - come si direbbe da queste parti "a babbo morto" - vuol dire che vengono commentati.

Con molta pacatezza: non c'è difficoltà a prenderne atto, ma questo è quanto stiamo votando. Noi abbiamo chiesto di sapere qual è il nostro intervento. Ci è stato detto che il Parlamento non deve saperlo e verrà informato

con la stessa pacatezza e anche con la speranza che si possa fare un passo in avanti - parlo in particolare al collega, senatore Romeo - prendiamo atto delle votazioni

Senatore Romeo, in queste ore, mentre qui discutiamo se il Governo italiano debba rendere un'informativa o una comunicazione tra due settimane, tutti gli si stanno esprimendo. C'è chi, come Erdogan, si schiera con Maduro e chi, come Bolsonaro, si schiera con la libertà dei cittadini venezuelani. Tutti i Governi si stanno esprimendo. L'Italia non si esprime perché questo argomento non è nel contratto di Governo?

Siamo qui. Perché non domani? Perché non domenica? In qualunque momento il Governo ha il dovere, meglio se con comunicazioni, di venire in questa sede a dirci se si schiera da una parte o dall'altra, perché non schierarsi oggi significa dare il via libera alla repressione sanguinosa di Maduro. Vogliamo capire o meno che due milioni di italiani rischiano la vita in quel Paese? Dobbiamo esprimerci subito. Il Governo deve scegliere da che parte stare. L'Italia sta con gli italiani in Venezuela.

abbiamo cioè fissato il principio che la politica estera è atemporale e che, in alternativa, le trivelle sono superiori per rilievo e importanza a due milioni di italiani che vivono in Venezuela. Questo principio è stravolgente, perché se la loro vita o quella di cittadini che votano per questo Parlamento è meno importante e quindi non porta in Aula il Ministro competente, fissiamo un criterio che non ha uguali nella storia, non della Repubblica italiana, ma dell'Italia unita, dal 1860 fino a questa mattina, ed è giusto che l'Assemblea lo sappia e si richiami ad una responsabilità che in centocinquanta anni in quest'Aula non è mai venuta meno, salvo nella giornata di oggi.

non è che l'ordine del giorno del Senato della Repubblica italiana viene prima di quello che accade nell'umanità. I liberi Parlamenti non possono determinare l'andamento della storia. Non mi illudo che se noi facciamo una discussione oggi, domani mattina o lunedì il mondo cambi, ma i liberi Parlamenti sono un presidio di libertà, per se stessi e per il mondo: questo stiamo dicendo in quest'Aula, quindi è opportuno parlare di quello che accade.

avere saggezza, poi si potrà discutere quando sarà, ma questo atteggiamento di mischiare i drammi della storia con la miseria delle trivelle e degli emendamenti è un errore che il Senato non può tollerare. Viva il Venezuela del popolo venezuelano! È questo che dobbiamo dire in questa sede oggi, perché c'è gente che rischia di andare sotto i carri armati e cosa verrà detto loro? Aspettate, sospendiamo la guerra civile, perché a Roma devono sapere quando ne parleranno? Non ci dobbiamo coprire di questa vergogna.

che il Venezuela, per fortuna, è stato considerato più importante di come ai miei tempi veniva considerato il Bangladesh. **Interventi su

il suo è un intervento di fine seduta. Ha tre minuti.

Guido Rossa era un operaio iscritto alla CGIL, un operaio militante del Partito Comunista Italiano, un operaio che non ebbe dubbi a schierarsi, a decidere da che parte stare e ad agire di conseguenza, anche in un momento storico - lo voglio ricordare - in cui lo scontro politico era tanto violento da mettere in gioco e a rischio la propria vita. un operaio e un sindacalista che lottava per la sua gente, per rendere più giuste e dignitose le condizioni di lavoro e quindi di vita, che credeva nella democrazia ed era pronto a battersi per difenderla da chi voleva annientare la Repubblica, colpendone i valori, gli spazi di convivenza democratica, il senso di comunità. Non ebbe dubbi a denunciare un collega di fabbrica dell'Italsider, che diffondeva volantini inneggianti alla lotta armata: Rossa fu il primo a farlo in questo Paese. Fece ciò che la sua coscienza gli indicò come giusto, quello che la sua comunità di riferimento, la CGIL, riteneva fosse una responsabilità di tutti i lavoratori per fermare i tentativi di infiltrazione brigatista nelle fabbriche e contrastare in ogni modo il terrorismo, che Luciano Lama definì nemico mortale della classe operaia. Come sapete, mai in CGIL ci furono atteggiamenti di comprensione verso quelli che qualcuno definiva «compagni che sbagliano»; mai ci fu un tentennamento di fronte a chi diceva di stare né con lo Stato, né con le BR. Non erano «compagni» quelli che uccidevano: non c'era nessuna altra parte dove i lavoratori e i sindacalisti potessero stare che non fosse quella dello Stato e della democrazia. Guido Rossa era fortemente convinto di questo, umanamente e politicamente; così convinto da agire, da rischiare, da non temere per la propria vita e per la propria famiglia; così convinto da essere scelto dai terroristi come uno di quelli che andava punito, colpito, ucciso. Quando Luciano Lama prese la parola nel giorno dei funerali, davanti a quasi 250.000 donne e uomini venuti a rendere omaggio a quell'operaio che aveva dato la vita per la democrazia, ribadì con fermezza la condanna di ogni forma di violenza e l'impegno del sindacato contro il terrorismo, a difesa della libertà e della Repubblica. Disse Luciano Lama: «Se il gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato, se (...) noi tutti (…) fossimo stati un solo grande testimone schierato contro il nemico della democrazia, forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata». Parole cui fecero eco quelle di un compagno di fabbrica di Guido, Paolo Perugino, dell'esecutivo del consiglio di fabbrica dell'Italsider: «Guido «Guido Rossa è stato ucciso perché non si è piegato, perché non ha ignorato, perché non ha avuto paura e ha voluto vivere fino in fondo, con coerenza, la sua scelta politica. Coloro che speravano, con questo assassinio, di chiuderci sgomenti nelle nostre fabbriche si sono sbagliati. Non sanno di quale ostinata rabbia e determinazione noi siamo capaci». Di quella mattina del 24 febbraio del 1979 e dei giorni successivi io ricordo personalmente, insieme a tanti altri, lo sgomento e l'infinita tristezza, certo, di un primo momento, ma poi la rabbia e la determinazione; la rabbia e la determinazione di tutto il movimento sindacale, di CGIL, CISL e UIL, e di tutto lo schieramento politico democratico che era stato vicino alle idee e alle battaglie di Guido. Per tutta l'Italia, quel giorno qualcosa cambiò, anche grazie a quella rabbia e a quella determinazione; la rabbia e la determinazione delle operaie e degli operai. Iniziò, così, la fine del terrorismo, che pur non risparmierà, purtroppo, altre vittime, ma che si ritrovò improvvisamente più isolato nelle sue deliranti rivendicazioni e nelle sue folli violenze. Ricordare oggi Guido Rossa qui significa, allora, ricordare e riaffermare il suo esempio e voglio con forza condannare le scritte apparse ieri, che sono un insulto non solo a lui, ma a tutta la memoria e a tutta l'Italia democratica della nostra storia. Ricordiamo Guido nell'anniversario del giorno in cui è stato ucciso, ma lo ricordiamo soprattutto per l'esempio della sua vita, per la forza morale, per il senso di giustizia e di uguaglianza, per lo spirito di solidarietà.

lo spirito di solidarietà, la generosità e il coraggio che l'hanno sempre caratterizzato, fino alla fine. Il suo non è, quindi, l'esempio di un martire, ma di un eroe civile. Certo, come ha ricordato ieri il presidente Mattarella nella cerimonia di ricordo a Genova, Guido non si proponeva di diventare un eroe, ma voleva essere fedele a se stesso, a ciò che intendeva costruire per il domani della sua famiglia, del quartiere in cui abitava, della fabbrica in cui lavorava, dell'intera società. «Non indugiò», sono ancora parole del Presidente, «a chiedersi se toccasse proprio a lui contrastare il terrorismo. Seppe però battersi per tutti». Ringraziare oggi oggi Guido Rossa e tutta la sua famiglia per quello che ha patito credo che sia un atto doveroso; lo ritengo giusto e un grande insegnamento per le giovani generazioni. Sono contenta che siano in Aula anche dei ragazzi che assistono Mi unisco, senza se e senza ma, al ricordo di Guido Rossa e lo faccio con un trasporto maggiore in quanto a me toccò essere presente ai funerali delle prime vittime delle Brigate Rosse, Giralucci e Mazzola, che vennero assassinati nella sede del Movimento Sociale Italiano a Padova. La mia solidarietà è quindi completa e vicina.

oggi stiamo andando contro tutte le regole sui tempi.

Fedeli e, anche da parte nostra, credo sia stato corretto e giusto ricordare quei tempi, anche sotto forma di insegnamento per il futuro, come è avvenuto oggi all'interno del Senato.

per associarmi, anche a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, al ricordo di questo lavoratore, sindacalista e cittadino che diventò, in uno dei momenti più drammatici del fenomeno terroristico, una riscossa autentica di cittadini comuni e lavoratori, che riaffermarono in quel momento il valore della democrazia e il rifiuto della violenza. Un saluto alla famiglia è doveroso, ricordando l'esempio fulgido di Guido Rossa, che è anche l'impegno di tutti i cittadini italiani per difendere i valori della democrazia e per fare in modo, se ce ne sarà occasione anche approfondendo il tema con dei dibattiti, perché sbornie di violenza, sbornie ideologiche di quel tipo non abbiano a ripetersi nel nostro Paese. *(Applausi).*

chiarezza, intendo ricordare a questa Assemblea e al Presidente che nel 2011 l'Agenzia delle dogane ha indetto un concorso per 69 posti per dirigente di seconda fascia. Di questo concorso si è parlato molto nelle aule dei tribunali amministrativi, ma soprattutto nelle Aule parlamentari, perché è un concorso che ha riportato molti vizi, a partire dalla correzione dei temi d'esame, che è stata svolta in modo personale da un membro della commissione e non in modo collegiale. Oltre a questo, sono successi degli scandali ben più gravi, tant'è che all'interno delle *Gazzette Ufficiali* che sono state distribuite durante il concorso vi erano le prove scritte svolte del concorso stesso, una cosa gravissima. Ne sono nate quindi indagini, anche di carattere penale, e il 1° febbraio ci sarà l'udienza davanti al giudice per le indagini Ebbene, ne sono susseguiti ricorsi, molti dei quali sono stati rigettati, ma in una sentenza di rigetto di uno di questi ricorsi si fa riferimento alla possibilità dell'Amministrazione di ritirare il concorso in autotutela. Poiché sono sicuro e certo di far parte di un Paese civile, civile, forse è il caso che questo concorso venga veramente ritirato, perché non possiamo avere il dubbio che alcuni possano passare questo concorso così pieno

In tema di rinnovabili, però, in Calabria si assiste ad una proliferazione abnorme di parchi eolici, complice la giunta Oliverio, naturalmente disposta a concedere VIA favorevoli e troppo spesso spalleggiata da certi dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali pronti, in materia di tutela del paesaggio, a chiudere anch'essi non uno, ma entrambi gli occhi. Per lo stesso motivo e con le stesse complicità, in una Regione che si spopola a ritmo serrato, la mamma delle discariche (siano esse per rifiuti del ciclo pubblico o speciali) è più prolifica della celebre scrofa bianca di Enea. Ciò mette a rischio la salute dei cittadini e attenta ai valori paesaggistici di un territorio di per sé votato invece all'agroalimentare di qualità e al turismo sostenibile. Non si può che solidarizzare, pertanto, con il gruppo Ambiente e Territorio di Mongrassano, nel Cosentino, oggi impegnato nella giusta battaglia contro l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Aria del vento, progettato dalla Gamesa energia Italia SpA (oggi Siemens Gamesa), contrastato dai residenti non per un rifiuto preconcetto della modernità, ma per ragioni sensate e condivisibili. Personalmente non finirò mai di deplorare la distorsione del linguaggio, per cui i nomi non rispecchiano più la sostanza delle cose: penso a «parco eolico» ma anche, nel campo del trattamento dei rifiuti, all'uso del termine «valorizzazione» per termovalorizzazione, cioè incenerimento, uso ormai talmente radicato che pure la tentata distruzione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese,

per interessare anche aree afferenti ai Comuni limitrofi di San Marco Argentano e Cervicati, alcune delle quali percorse dal fuoco negli anni scorsi. Ebbene, è notorio che detta dorsale è attraversata da un'importante frattura della crosta terrestre: la faglia San Fili-San Marco Argentano. Non basta, perché l'intera macroarea denominata Catena costiera e fascia pedemontana, come si legge nell'aggiornamento del programma di previsione e di prevenzione dei rischi e del piano di emergenza della Provincia di Cosenza, adottato nel 2014, si caratterizza anche per un elevatissimo rischio di frana. Abbiamo ancora tutti negli occhi la cancellazione dell'abitato e le gravi conseguenze per tutto il circondario causate dalla frana che ha interessato la vicina frazione Cavallerizzo del Comune di Cerzeto. In un territorio così fragile dal punto di vista geologico, il parco eolico Aria del vento si segnala negativamente anche sul piano ambientale, sia per il mancato rispetto delle distanze prescritte dalle più vicine aree naturali protette della rete Natura 2000, sia per la coincidenza con uno dei sentieri di crinale inseriti dalla Regione Calabria nel progetto di valorizzazione...

le vicende che riguardavano il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, che da vent'anni il territorio della Provincia di Cuneo chiede, dato che la città di Cuneo è ancora l'unico capoluogo di Provincia in Italia non collegata ad un'autostrada. fine della passata legislatura, il ministro Delrio aveva concordato un *cross financing* autorizzato dall'Unione europea, per il quale a fronte di un prolungamento di concessione di quattro anni della Torino-Milano, la società concessionaria avrebbe realizzato questo completamento. Il nuovo ministro Toninelli aveva chiesto di poter esaminare le carte per fare una valutazione e a gennaio di quest'anno una deputata del MoVimento 5 Stelle ha rilasciato una dichiarazione, nella quale ha detto che la porta del Ministro era sempre aperta e se qualcuno avesse voluto parlare col Ministro

di sospendere tutto il percorso fatto e di fare sì il completamento, ma con fondi dello Stato. Sono quindi qui a sollecitare la risposta all'interrogazione (e nella giornata di ieri ne abbiamo presentata una ulteriore, alla luce dei nuovi elementi sopraggiunti), ma soprattutto a chiedere che il Governo ci dica cosa intende fare. Sotto questo profilo, ho sentito il ministro Toninelli dire che rifaranno tutti gli accordi, perché li faranno decisamente migliori e maggiormente nell'interesse del territorio e delle comunità.

di spesa pubblica e non fare l'accordo di *cross financing*, la menassimo altri due anni, con un costo di qualche centinaia di milioni di euro per l'economia del territorio. Non capiamo quale possa essere la logica che sta dietro a quest'approccio folle

Signor Presidente, intervengo con riferimento anche al dibattito sul Venezuela per sollecitare ancora una volta, la costituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, che solo in questa legislatura e solo in questo ramo del Parlamento non è ancora stato ricostituito. Si sono citati gli italiani che vivono in Venezuela, che sono in grande numero: ebbene, il luogo deputato istituzionalmente per approfondire e avanzare proposte relative a tali tematiche è il Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

audire quindi il sottosegretario Merlo sulla situazione specifica degli italiani in Venezuela? Potrebbe essere opportuno. *(Applausi